con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato la sig.ra Valentina VEZZALI a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. F.to Mario Draghi».

recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale provvedi- mento, all’articolo 18, abroga tutta una serie di norme che hanno a che fare con il controllo della qualità alimentare. Tra queste, viene abrogata anche

il rischio che prodotti in parte in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti, adulterate o contraffatte, colorate artificialmente - e tutta una serie di altre casistiche casistiche minanti la salute umana - non ricevano più alcuna multa perché tra il reato grave e il nulla è stata abolita tutta la fattispecie dei comportamenti colposi intermedi.

giorno: Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e del 26 marzo 2021